offrire al paziente una dignitosa qualità della vita attraverso un'assistenza che varia in base ai bisogni del paziente e della sua famiglia. Questa legge interessa 250.000 persone che ogni anno si trovano in queste condizioni, tra le quali 11.000 bambini. Di queste, 160.000 sono malati terminali e la restante parte sono pazienti con patologie croniche, cardiache, respiratorie, neurologiche, metaboliche e anche infettive. L'universo del malato terminale apre una serie di problematiche. È evidente infatti che la domanda di cura che ogni paziente rivolge al medico tende a differenziarsi in maniera sostanziale a seconda della malattia e del livello di sofferenza che provoca in lui e nella sua famiglia, ma anche a seconda degli stili di vita, dei suoi valori e della sua personalità. Tutta la legge tende a mettere al centro dell'attenzione non la malattia, ma il paziente con tutti i suoi bisogni. È limitativo infatti parlare solo di dolore fisico o di terapia farmacologica. Il malato, soprattutto oncologico, manifesta una serie di bisogni fisici, funzionali, psicologici, esistenziali e sociali che vanno riconosciuti e affrontati nella loro complessità, specie nelle fasi avanzate-terminali, dove la sofferenza è totale e non solo fisica. Tanto che, non a caso, alle terapie farmacologiche è associata la possibilità di un sostegno psicologico, spirituale e sociale rivolto sia alla persona malata che, cosa cosa importante, alla sua famiglia, a quella famiglia che rappresenta ancora oggi in Italia l'ammortizzatore sociale più importante di cui disponiamo. disponiamo. È positiva la particolare rilevanza che si è data a quelle strutture che ospitano i minori, così come i soggetti diversamente abili, che alla loro condizione persistente associano una condizione nuova ancora peggiore. Mai come in questi casi la medicina può dimostrare il suo volto umano e l'attenzione per la dignità del vivere e del morire. Secondo il testo, l'accesso alle prestazioni erogate dalla rete di cure palliative e dalla rete delle terapie contro il dolore è regolato dai principi generali dell'universalità, dell'equità e dell'appropriatezza. In modo corretto, si identificano due reti separate, una per le cure palliative e una per la terapia del dolore, facenti capo ad un'unica struttura dipartimentale, per agevolare la necessaria attività di coordinamento. Il circuito virtuoso della rete è composto dalla struttura ospedaliera, nei momenti di particolare criticità clinica, dall'*hospice*, cioè ospedale senza dolore, come luogo di accoglienza, e infine la propria la propria abitazione (*home*), dove stare il più a lungo possibile godendo di tutte le cure di una buona assistenza domiciliare. Fanno parte della rete anche il medico di famiglia, i pediatri di libera scelta, un centro di telemedicina, la farmacia distrettuale e ospedaliera. Detto questo, qualche cosa ci preoccupa vedendo i dati; faccio l'esempio del censimento degli *hospice*: 51 si trovano in Lombardia, 5 in Campania e 15 nel Lazio. Questo dato ci pone davanti il problema delle difformità regionali, quindi il rispetto del criterio di equità. Molte Regioni svantaggiate non sono in grado di assicurare un'assistenza domiciliare adeguata; non tutte le Regioni hanno concluso il sistema di accreditamento, per cui manca la possibilità di creare un unico modello nazionale della rete in considerazione dell'autonomia regionale.

prevedere una serie di sanzioni per quelle Regioni che fossero inadempienti o usassero le risorse che noi proponiamo in questa legge per altri scopi. Naturalmente, in questo criterio di equità regionale rientra anche la formazione del personale impegnato nelle due reti. È indispensabile infatti costituire dei percorsi formativi di tipo interdisciplinare multiprofessionale. Altra parte importante è rappresentata dalla necessità di informare i pazienti e le loro famiglie; infatti, purtroppo, solo il 60 per cento dei pazienti terminali e quasi tutti quelli che non hanno una malattia oncologica sfuggono oggi alla rete delle cure palliative. Ecco perché è necessaria una campagna di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e dell'applicazione della terapia del dolore. Nel provvedimento è poi prevista una semplificazione, che non vuol essere una liberalizzazione, per l'impiego delle sostanze stupefacenti a scopo sanitario. Sparirà il ricettario speciale per la prescrizione degli oppioidi. Il livello del dolore - credo che questo sia un aspetto importante - sarà costantemente monitorato nelle corsie degli ospedali; medici e infermieri dovranno costantemente riportarlo nella cartella clinica.

Noi speriamo che questa buona legge non rimanga un contenitore quasi vuoto, senza finanziamenti confacenti, e che sia fatto uno sforzo adeguato perché i bisogni di questi pazienti sono i bisogni di tante famiglie italiane.

Signor Presidente, colleghi, il voto dell'Italia dei Valori su questo disegno di legge sarà un voto decisamente favorevole.

ringrazio anch'io il relatore, il collega De Lillo, per l'ottima capacità di sintesi, dal momento che questo testo, non dimentichiamolo,

di altri colleghi dell'opposizione. È quindi un testo che proviene da una sintesi di culture, di sensibilità, di esperienze diverse.

che abbiamo assolto a tutto il nostro dovere, e quindi chiuderci in una sorta di autoreferenzialità pensando di poter stare a posto con la nostra coscienza.

tanti pazienti e cittadini che hanno bisogno di accedere alla medicina palliativa e alla terapia del dolore. I numeri sono già stati abbondantemente ricordati in Aula in più occasioni:

si trovano spesso sole, abbandonate di fronte ai delicati risvolti affettivi e psicologici che comporta la cura di un malato terminale.

È un atto di civiltà perché il nostro Paese è tra i più arretrati in Europa rispetto alle garanzie di accesso alla medicina palliativa e alla terapia del dolore.

ma sono anche espressione di un diritto fondamentale: quello del rispetto della dignità della persona anche nei momenti più delicati. delicati. Il secondo errore che possiamo commettere è quello di pensare - e sul punto vorrei che ci fosse un po' di attenzione da parte di tutti

Dico questo perché, nel nostro sistema legislativo, di provvedimenti e di disposizioni legislative sulla materia ne avevamo già tantissimi e da moltissimi anni. Nel 2001 un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aveva già stabilito che l'assistenza domiciliare e quella residenziale e ambulatoriale nei confronti dei malati terminali

Per non parlare poi della legge n. 39 del 1999 dell'allora ministro Bindi: anche quella era una legge che conteneva disposizioni sulla realizzazione di una rete di *hospice* nel nostro Paese. allora che non ha funzionato? Di *hospice*, sia pure pochi, sia pure in maniera disomogenea e disarticolata tra Nord e Sud, ne sono stati realizzati (gli ultimi dati del Ministero parlano di circa 126 *hospice,* di cui un'ottantina realizzati con fondi statali e il resto con fondi di diversa fonte, tra cui privati). di diversa fonte, tra cui privati). Non ha funzionato una cabina di regia, anche a livello regionale, che creasse realmente una rete, una continuità di percorso assistenziale, tant'è che questi *hospice* sono diventati quasi dei punti di riferimento isolati rispetto ai bisogni e alla richiesta di assistenza dei pazienti. Ed allora, non basta semplicemente un provvedimento di legge di legge per poter dire che potremo successivamente passare con tranquillità all'attuazione dei dispositivi importanti che in esso sono contenuti. Vedete, questa legge contiene due aspetti molto significativi. luogo, si stabilisce il diritto alla continuità assistenziale, cioè un percorso che dia la possibilità di integrare l'attività degli ospedali con quella degli *hospice* e delle residenze e con l'assistenza domiciliare. Il secondo diritto che viene stabilito in questa legge è la libertà del paziente di scegliere il luogo dove farsi curare, ma soprattutto dove poter vivere gli ultimi giorni della sua vita. Vorrei rivolgermi in modo particolare al rappresentante del Governo che avrà su di sé grandi responsabilità: nel nostro Paese, signor Ministro, il 75 per cento degli italiani che vivono questa situazione drammatica chiede di poter completare gli ultimi giorni della vita nella propria abitazione. Questa sensibilità va colta nella misura in cui sarà necessario, rispetto ad una rete di *hospice*, potenziare soprattutto l'assistenza domiciliare

Il mio intervento sarà impostato in maniera molto diversa. Per la prima volta il Parlamento si occupa degli esclusi e degli emarginati;

vi sono già i primi sintomi: l'assistenza ai malati terminali potrebbe essere inserita in quegli scandali generali che attraversano la sanità italiana. Bisogna recuperare il concetto di fondo,

però non è stata detta, signor Ministro, e ci tengo a dirla perché credo sia il punto centrale della cura del dolore e delle cure palliative. Mi riferisco all'integrazione socio-sanitaria.

L'ammalato e la famiglia non possono assistere a sceneggiate su deleghe di responsabilità al Comune, alla ASL o altrove.

importa se è a carico del Comune, della ASL o di altri. Questa è la grande rivoluzione che dobbiamo portare avanti, ossia l'integrazione: da anni ne parliamo, ma non ci riusciamo.

Mi dispiace che sia stato soppresso l'articolo recante le misure di penalizzazione delle Regioni inadempienti. Inventiamo qualche altra cosa, ma è importante che si tolga questo steccato tra Regioni. Regionalizzare è un bene,

perché si notano dei punti di negatività e delle proposte, magari sottovoce, in cui si vuole andare a mio parere troppo verso il privato.

un vuoto quasi ventennale, un giorno che gli operatori del settore e soprattutto un grande stuolo di pazienti stanno aspettando da tantissimi anni; eppure credo che in questa giornata non sia il caso di utilizzare toni trionfalistici,

che giocoforza ha dovuto limitare i fondi a disposizione per questo disegno di legge, rendendolo da questo punto di vista probabilmente un incompiuto, un qualcosa che non dà una completa risposta e una completa soddisfazione

Il grosso rischio è che questa legge possa mantenere nettamente separate le due reti: la rete delle cure palliative rispetto alla rete della terapia del dolore. È sicuramente vero che andare incontro ha bisogno sia di cure palliative che di terapia del dolore: questa legge è imperniata infatti prevalentemente sul malato terminale, sul malato oncologico, e a questo riesce sicuramente a dare un'ottima risposta. Grazie a questa legge si auspica che si andrà a completare in maniera fattiva la rete degli *hospice* e quindi si riuscirà davvero ad implementare, a livello territoriale e ospedaliero, ospedaliero, l'assistenza al malato terminale prevalentemente oncologico. Resta però scoperta o comunque rischia di rimanere figlia di un Dio minore tutta la parte dedicata alla terapia del dolore *tout court*. Non dimentichiamoci, infatti, che non esiste solo il dolore oncologico del paziente terminale, ma esiste anche il dolore cosiddetto cronico-benigno: penso al dolore neuropatico, al dolore vascolare e a tanti altri dolori che sono addirittura peggiori rispetto a quello oncologico, avendo una durata nel tempo notevolmente più lunga e creando limitazioni

fondamentalmente per quel limite economico - siamo dovuti passare sotto le forche caudine del bilancio per riuscire ad approvarla - e quindi le risorse non sono sufficienti per riuscire a coprire a 360 gradi tutte le richieste. In particolar modo, non sarà possibile mettere assieme l'offerta delle due reti delle cure palliative e della terapia del dolore. Questo è il grosso limite della legge, ma è anche la grande occasione che essa ci offre. Come Lega Nord non possiamo che essere favorevoli e vedere molto bene questa possibile evoluzione: di fatto, è la prima volta che ci troviamo di fronte ad una legge delega in senso federalista della materia, e

la possibilità di stanziare risorse proprie, di interpretare tutto ciò che questa buona legge - lo ripeto - dà loro come possibilità per riuscire a mettere in campo soluzioni vincenti per i propri cittadini. Parlandone in questi giorni con il ministro Fazio e conoscendo la sua serietà e professionalità, non ho dubbi che riuscirà in questo intento. Nella Conferenza Stato-Regioni, il compito del Ministero e dell'istituzione nazionale sarà proprio quello di spronare le Regioni a completare la gamma di offerta in maniera tale che si possa avere una copertura contro il dolore e a favore delle cure palliative su tutto il territorio nazionale. Rimane il rammarico - lo raccontava anche ieri il collega Mascitelli - che a questa legge sia stato riconosciuto un quinto degli stanziamenti riservati al Comune di Catania e un decimo degli stanziamenti dati al Comune di Roma. Non è sicuramente un buon auspicio. Se dovessimo utilizzare il vecchio proverbio «chi ben comincia è a metà dell'opera», cominciamo veramente molto male. Auspico, però, che in sede di Conferenza Stato-Regioni e soprattutto per l'autoresponsabilizzazione delle Regioni stesse, mettendole anche in competizione l'una con l'altra per fare bella figura, si possa davvero riuscire a dare una risposta concreta a questo tipo di problema. intervento ringraziando tutti i colleghi della Commissione, a partire dal suo Presidente, e soprattutto il relatore De Lillo che è sapientemente riuscito a mettere assieme un testo particolarmente complesso, nonché il Governo e il ministro Fazio in particolare, quale ci è stato molto vicino. Licenziamo oggi questo provvedimento - credo - con il massimo sforzo che potesse essere fatto dal Senato per sistemare alcune imperfezioni che ci sono giunte dalla Camera e per offrire alle Regioni una possibilità di lavoro veramente concreta.

Innanzitutto rivolgo un ringraziamento non rituale ai colleghi della Commissione, al relatore De Lillo, al presidente Tomassini e al Ministro il quale, senza grandi discorsi ma con i fatti, si è dimostrato estremamente collaborativo nella relazione con il Parlamento per poter migliorare il disegno di legge

E allora ieri qualcosa in più si poteva fare. Fermarci di fronte a fatti tecnici non sempre è positivo, anzi in questo caso ritengo sia stato estremamente limitativo e non soddisfacente. Questo è il mio più grande rammarico. Certo, alla fine comunque la soddisfazione prevale. Innanzitutto perché si tratta di una legge di iniziativa parlamentare, uscita condivisa dalla Camera e condivisa anche qui: segno che il Parlamento può operare bene

euro sono stati buttati via, e non troviamo magari qualche decina di migliaia di euro per pagare le ricette ai pazienti e ai malati e per sostenere finanziariamente i provvedimenti sul rischio clinico e le malattie rare. Penso che su questo dobbiamo fare una riflessione.

hanno interpretato il segno di un tempo che stava cambiando: la tecnica medica ci portava avanti, la cronicità diventava un problema nel Paese, questi pazienti non potevano essere abbandonati a se stessi e bisognava seguirli, negli ospedali, a domicilio,

in esame noi affermiamo il diritto alle cure, il libero accesso e la semplificazione terapeutica, il rispetto della dignità umana, dell'uomo malato e, soprattutto, malato nella sua fase terminale, quando soffre di più. Sanciamo il no all'abbandono terapeutico, evitando però l'accanimento e garantendo a tutti il sostegno vitale

la seconda tappa di un percorso legislativo ampio, iniziato con l'approvazione della legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Credo che da tutti noi, anche dai non addetti ai lavori, che l'approvazione del provvedimento sulle cure palliative e sulla terapia del dolore rappresenta per certi versi l'altra faccia della luna: entrambi si pongono un unico obiettivo; entrambi i provvedimenti mostrano che il Parlamento ha deciso in modo coerente e in modo fattivo di prendersi cura delle gravi disabilità, del fine vita, del dolore, del disagio e della sofferenza che spesso accompagnano l'ultimo tratto della nostra esistenza. Se da una parte abbiamo voluto ribadire con la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento il nostro rifiuto all'eutanasia, all'accanimento terapeutico, al suicidio assistito, ed affermare dall'altra con chiarezza che una vita umana conserva la sua piena dignità anche se vive in condizioni di sofferenza e di grave disabilità, non avremmo certo potuto lasciare il malato e la famiglia soli e abbandonati alle loro difficoltà, ai loro disagi, al loro dolore. La risposta del Parlamento sarebbe stata monca e incongruente; non c'è dubbio infatti che una buona rete di cure palliative e di terapie antalgiche non solo aiuta a controllare il dolore e la sofferenza del malato nella molteplicità delle sue manifestazioni, ma aiuta anche a superare quel rischioso senso di abbandono che può cogliere il malato sofferente e a prevenire così i momenti di crisi e possibili forme anche di richieste eutanasiche. Consentitemi perciò innanzitutto e brevemente di riconoscere ai deputati di avere svolto un lavoro egregio, conclusosi con l'approvazione *bipartisan* e unamime del provvedimento che ci apprestiamo a votare questa mattina, e di testimoniare altresì che la Commissione igiene e sanità del Senato, il suo presidente, senatore Tomassini, e il relatore al provvedimento, senatore De Lillo, in collaborazione con il ministro Fazio, hanno lavorato con attenzione e con il contributo prezioso di tutti i partiti, apportando miglioramenti ma senza intaccare i principi di fondo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati. Il testo di oggi avvicina lo Stato al malato cronico, al malato sofferente, al malato terminale, che oggi, purtroppo, in assenza di una legge, non può contare né su una rete per le cure palliative né su un percorso chiaro per la terapia del dolore. attualmente non è in grado di incontrare strutture di assistenza, ad eccezione di pochi centri situati prevalentemente nel Nord del Paese. Allorché questo provvedimento potrà diventare legge, migliaia di pazienti con patologie croniche o dolorose e circa 250.000 pazienti in fase terminale di cui 150.000 affetti da patologia oncologica - sentiranno finalmente la presenza del Servizio sanitario nazionale e si sentiranno meno soli. Accennavo poc'anzi all'esistenza fino ad oggi di pochi centri specializzati e prevalentemente nel Nord d'Italia: una differenziazione geografica, quella tra il Settentrione e il Mezzogiorno, insopportabile, che viola il principio dell'uguaglianza dei diritti e in particolare del diritto alla salute che deve rimanere assoluto e a valere per tutti noi. È per questo che il provvedimento, pur nel rispetto delle autonomie regionali, prevede che spetti al Ministero della salute una funzione di controllo e di coordinamento sulla rete delle cure palliative e della terapia del dolore: si tratta di funzioni fondamentali per garantire un'assistenza omogenea sul territorio, ma anche per raggiungere *(Brusìo).* Da oggi, su tutto il territorio nazionale, il paziente terminale sarà assistito, a seconda delle esigenze e delle condizioni cliniche, a casa, in *day hospital*, in ambulatorio, in ospedale e in *hospice*, senza essere costretto a vagare da una struttura sanitaria all'altra. Certamente, uno degli aspetti più rilevanti del testo è che con l'istituzione di due reti, quella delle cure palliative e quella della terapia del dolore tra loro coordinate, si raggiungono i due risultati di cui parlavamo. Sono presenti gli studenti dell'istituto di istruzione superiore «Luigi Einaudi» di Canosa di Puglia, in

Dicevamo che uno degli aspetti più rilevanti del testo è che con l'istituzione delle due reti, quella delle cure palliative e quella della terapia del dolore, tra loro coordinate, si raggiungono due risultati: da una parte riporta, attraverso la rete nazionale, la responsabilità centrale dell'indirizzo del sistema sanitario nazionale, anche nell'attuazione delle singole Regioni, al Ministero; dall'altra, riuscirà a garantire la continuità assistenziale del malato dall'ospedale al suo domicilio in tutte le fasi della malattia. La costituzione di *hospice*, servizi di assistenza domiciliare e centri di assistenza specialistica di terapia del dolore, con un percorso preordinato sulle esigenze cliniche del paziente, comporta un cambio sostanziale in uno dei settori più importanti e delicati dell'assistenza sanitaria, portando il paziente, e non più la struttura, al centro del sistema di assistenza. Sono convinto che solo così noi porremo fine ai disagi del paziente e della famiglia e anche agli sprechi di denaro pubblico e mostreremo, finalmente, il volto umano dell'assistenza sanitaria. Ma, cari colleghi, nulla si fa, né si può immaginare di modificare, senza un'adeguata formazione degli operatori sanitari. Va pertanto dato merito al disegno di legge che stiamo per votare di aver previsto percorsi didattici specifici ed omogenei su tutto il territorio, perché gli enormi e continui progressi della medicina richiedono che il sistema sanitario, le università e le società scientifiche si adeguino, colmando quanto prima il ritardo nella formazione di questi particolari settori. Nulla si riesce a fare senza una campagna di informazione istituzionale che dia notizia al cittadino della possibilità di usufruire di queste nuove realtà. Non si tratta soltanto di informare i cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni e neppure soltanto di coinvolgere i medici di medicina generale, finora purtroppo restii e timorosi nei confronti della terapia del dolore. Si tratta, invece, di rendere consapevole l'opinione pubblica che può contare su un'efficiente rete di terapia del dolore e delle cure palliative. Signor Presidente, non occorre essere medici o operatori sanitari per comprendere l'importanza della semplificazione delle procedure, che in questo disegno di legge abbiamo ottenuto con chiarezza. Il disegno di legge prevede che la prescrizione di farmaci antidolorifici, attraverso l'utilizzo del ricettario del Servizio sanitario nazionale, superi le difficoltà presenti nella normativa attuale. Sono la medicina e la scienza, nella loro continua evoluzione, a chiederci di andare incontro al bisogno del malato, di scavalcare un inutile e dannoso *iter* burocratico che richiedeva bolli, copie e trafile varie. Colleghi, questa varie. Colleghi, questa è senz'altro una legge buona, che non può dividere, che non abbisogna di grande prove di dialogo tra maggioranza ed opposizione, perché tutti noi siamo uniti nella speranza di poter dare un sollievo a chi vive nel dolore. Pertanto, auspichiamo di licenziare il testo all'unanimità, reiterando quanto già avvenuto alla Camera. Un'unanimità che sarebbe senz'altro un segno di grande civiltà e un messaggio di speranza per il Paese.

è un privilegio e un onore aver seguito, prima alla Camera e poi al Senato, l'*iter* di questo disegno vorrei segnalare un aspetto. Ho osservato che è stato rilevato, dall'opposizione ma anche dalla maggioranza, che forse si poteva fare di più.

sede di Conferenza Stato-Regioni, l'attuazione piena della legge in tutte le Regioni nell'ambito dei LEA e a promuovere, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, se necessario, l'iniziativa a destinare risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale. Infine, il Governo si impegna affinché la relazione annuale alle Camere non sia un atto formale ma una reale verifica dell'implementazione delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative nel nostro Paese.

nella Conferenza dei Capigruppo di ieri si sono stabiliti i tempi per la discussione del decreto milleproroghe, sul quale però sono stati presentati 650 emendamenti,

Quindi chiedo a lei, signor Presidente, di trasmettere al presidente Schifani la richiesta del nostro Gruppo di un'ulteriore fissazione dei tempi, perché con le due ore a disposizione del mio Gruppo non si può affrontare con l'approfondimento e con la compiutezza necessarie

Presidente, colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori si associa alla richiesta del Gruppo del Partito Democratico.

Signor Presidente, concordo con la presidente Finocchiaro e con il presidente Belisario. Mi permetto di sottolineare che quello che sta capitando sul decreto milleproroghe non è altro che l'effetto della finanziaria *light* o presunta tale. La maggioranza si è vantata di aver fatto una finanziaria semplice, con quattro norme essenziali, intelligibili, chiare e così via. La verità è che, con

con norme quali la proroga dello scudo fiscale, con norme che riguardano il reclutamento del personale la pubblica amministrazione, con norme che riguardano la reintroduzione dell'esenzione fiscale sul tartufo. Insomma, con tutto uno zibaldone di norme che non credo abbiano nulla a che vedere con la stretta interpretazione delle disposizioni che riguardano la proroga di alcuni termini la cui scadenza può pregiudicare seriamente l'andamento di una serie di attività delle amministrazioni dello Stato. Il tema è questo. Allora, o la Presidenza utilizza i poteri che le sono conferiti dal Regolamento sotto il profilo delle censure di inammissibilità degli emendamenti e impone una regola che consenta al al Parlamento, al Senato e alla Commissione di concentrarsi solo ed esclusivamente su quelle poche ed essenziali disposizioni che riguardano la proroga dei termini rispetto alle quali vi è

che ridisciplina e riforma sostanzialmente le procedure per l'approvazione del bilancio dello Stato e delle disposizioni finanziarie, e che dovremo esaminare alcune di queste norme, che sono state inserite o che verranno inserite in Commissione nel milleproroghe, senza avere un quadro dei collegati ordinamentali in cui naturalmente queste norme dovrebbero andare. È un modo di procedere che non ci può trovare d'accordo, perché non ci mette nelle condizioni di lavorare seriamente.

Signor Presidente, apriamo un dibattito sulla cosiddetta legge comunitaria che ci illudiamo - almeno noi che ci occupiamo di questa materia - possa indicare qualche sentiero nuovo, qualche idea innovativa per trattare questa complessa materia, soprattutto quest'anno, in un anno in cui la legge comunitaria si colloca in una fase di sensibili innovazioni per la cornice europea. Innanzitutto, è la prima

dei membri della Commissione europea, con la grande riforma del Consiglio europeo, con un Presidente destinato a durare due anni e mezzo e con un Ministro degli esteri, che finalmente si può definire tale, quindi dotato di competenze reali. L'aspetto routinario della legge comunitaria, quindi, ne esce nobilitato, anche se siamo di fronte ad una seconda lettura. Prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, occorre ricordare che, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento del Senato, l'annuale disegno di legge comunitaria deve essere esaminato congiuntamente alla Relazione annuale grazie 144-*bis* del Regolamento, oggi noi ci troviamo ad esaminare, insieme al disegno di legge comunitaria 2009, anche la Relazione annuale relativa al 2008, sebbene solo alla fine dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale problematica temporale, unitamente alla considerazione della diversa natura dei due atti (meglio ricordare che la Relazione è più di carattere politico-programmatico e più attinente

abbinando l'esame della Relazione annuale all'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Consiglio. A tale riguardo si ricorda che nel febbraio scorso è stato trasmesso alla Presidenza del Senato un documento contenente alcune proposte di modifica regolamentare, a firma di tutti i membri della 14a Commissione, nel quale si propone tra l'altro una modifica all'articolo 144-*bis* del Regolamento, appunto nel senso di prevedere un esame disgiunto del disegno di legge comunitaria rispetto alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

è una seconda questione, oggetto delle proposte di modifica, che riguarda la competenza della 14a Commissione sui provvedimenti *ex* articolo 10 della legge n. 11 del 2005, la cosiddetta legge Buttiglione, che prevede la possibilità di adottare dei «provvedimenti anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso». La proposta di modifica regolamentare va nel senso di prevedere che quei provvedimenti di contenuto analogo a quello della legge comunitaria che siano finalizzati alla necessaria attuazione di obblighi comunitari siano anch'essi esaminati

Peraltro, si è consolidata negli ultimi anni una prassi di cui l'ultimo esempio è il cosiddetto decreto salva-infrazioni, il decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135, approvato dal Senato in prima lettura il 4 novembre. A tale riguardo, ritengo opportuno accennare ad una problematica di carattere ordinamentale emersa durante l'esame del citato decreto‑legge. Mi riferisco al cosiddetto oggetto proprio della legge comunitaria, in base al quale il contenuto di tale provvedimento deve essere limitato

è spesso accaduto che il disegno di legge presentato dal Governo contenesse *ab origine* disposizioni che non rispondevano a tale necessità. A tale riguardo, mentre il Regolamento consente di effettuare un vaglio di ammissibilità per estraneità di materia sugli emendamenti, lo stesso non è previsto anche per il testo del disegno di legge, che quindi, in passato, è giunto all'approvazione definitiva contenendo norme non rispondenti al criterio dell'oggetto proprio della legge comunitaria. Insomma, si è realizzato puntualmente il famoso *omnibus*, sul quale ognuno caricava tutto e il contrario di tutto, magari recuperando qualche norma rimasta esclusa dalla legge finanziaria. Tengo a precisare che questa mia osservazione, che ritengo del tutto pregnante nell'attuale congiuntura parlamentare, assume un valore squisitamente tecnico-politico, in quanto si riferisce ad un *modus operandi* fatto proprio negli ultimi anni da Governi di diverso orientamento politico, quindi sia di centrodestra sia di centrosinistra. Una spinta ulteriore a trovare proposte capaci di semplificare ed accelerare la procedura deriva dall'applicazione del citato Trattato di Lisbona e dal più incisivo ruolo che esso assegna ai Parlamenti nazionali, soprattutto nella fase ascendente della formazione delle normative comunitarie. Passiamo molto rapidamente all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2009. Occorre ricordare che esso è stato presentato presso l'altro ramo del Parlamento il 19 maggio scorso e conteneva solo nove articoli. Oggi, all'esame di

quelli che appaiono più rilevanti, raggruppandoli per argomenti, per categorie tematiche. Una prima categoria è quella contenente le disposizioni ordinamentali di modifica della legge n. 11 del 2005, la nostra legge quadro, che disciplina il rapporto tra l'Italia e l'Unione europea. Con l'articolo 6 del disegno di legge approvato dalla 14a Commissione del Senato si modifica l'articolo 2 della legge n. 11 del 2005, relativo ai compiti del CIACE (Comitato a tener conto dei pareri espressi dal Parlamento nell'ambito dell'elaborazione delle linee politiche dell'Esecutivo relative alla fase ascendente del processo legislativo europeo. Analogamente, con l'articolo 7 approvato dalla Camera dei deputati si introduce nella legge n. 11 un nuovo articolo, che obbliga il Governo a tener conto degli atti di indirizzo emanati dalle Camere in fase ascendente, nell'ambito dei suoi rapporti con le istituzioni comunitarie. Queste due disposizioni sono dunque dirette ad un rafforzamento del ruolo del Parlamento nella fase ascendente del processo legislativo comunitario, anche in considerazione dell'accresciuto ruolo, come si è detto, attribuito dal Trattato di Lisbona Lo stesso articolo 7 obbliga il Governo ad assicurare la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere per predisporre i programmi nazionali di riforma nell'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. L'ultima parte dell'articolo 7, relativa alle informative al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso, prevede che il Governo, in relazione a specifici atti o procedure di infrazione, trasmetta tempestivamente tempestivamente - è enfatizzato questo avverbio - alle Camere, su loro richiesta o in casi di urgenza, non solo le informazioni - questa è una novità - ma anche i documenti anche i documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere. Ciò significa che la trasmissione degli atti delle procedure di infrazione acquisirebbe con questa norma una base giuridica legislativa. Tale disposizione è stata estesa, grazie ad un emendamento approvato dalla 14a Commissione del Senato, anche alle procedure di infrazione che sono alla base di disposizioni legislative del Governo sottoposte all'approvazione del Parlamento. In tali casi, infatti, la nuova disposizione richiede che il Governo comunichi al Parlamento non solo le relative informazioni ma anche i relativi documenti più significativi. La 14a Commissione del Senato, inoltre, ha ritenuto opportuno precisare che la trasmissione al Parlamento delle informazioni e dei documenti relativi alle procedure di infrazione possa avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 19, ovvero anche secondo modalità informatiche, informatiche, nonché che il Governo possa raccomandarne l'uso riservato. In merito alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevista dall'articolo 15 della legge n. 11 l'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, affianca ad essa una nuova relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre e contenente le linee programmatiche che il Governo propone per l'anno successivo. Questa nuova relazione programmatica rappresenta quindi un punto di sintesi importante per lo svolgimento di un approfondito dibattito parlamentare sulla politica europea italiana. In riferimento invece alla consueta Relazione annuale sull'anno pregresso, c'è una novità importante che proponiamo come Commissione all'attenzione del Senato; potremmo essere gli apripista di una riforma che da tempo molti proponevano per recuperare un *handicap* denunciato inutilmente e che in questa comunitaria potremmo con il vostro voto anche colmare. In merito alla consueta Relazione annuale la Commissione ha approvato un emendamento che ne integra e precisa i contenuti, prevedendo che il Governo riferisca specificamente anche in merito ai lavori svolti presso il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, nelle sue diverse formazioni,

del principio di sussidiarietà che, sulla base del Trattato di Lisbona, viene applicato in tutti gli Stati. Si tratta dell'articolo 9 del disegno di legge che, in vista della futura riforma della legge n. 11, introduce un principio fondamentale in relazione ai rapporti tra Governo e Parlamento nella fase ascendente. Nello spirito di una leale collaborazione tra l'Esecutivo e il *côté* parlamentare, si chiede al Governo di fornire, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di un progetto di atto legislativo europeo, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi a questo progetto, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito. In particolare, tale informazione, che potrà essere fornita anche in forma scritta, dovrà contenere una valutazione complessiva del progetto europeo, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie opportune modifiche; dovrà evidenziarne l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese; dovrà contenere una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno. Anche in tale contesto, la 14a Commissione ha ritenuto di consentire al Governo di raccomandare l'uso

disposizioni concernenti singoli settori che necessitano di un adeguamento per risolvere procedure di infrazione o comunque per rispondere ad esigenze derivanti dall'ordinamento comunitario. A tale riguardo non posso non citare un tema ormai annoso, quasi oggetto di un abbonamento, che rischia di diventare cronico se non viene risolto in questa sede, dell'adeguamento della legislazione italiana alla normativa europea in tema di gestione della caccia in rapporto alla tutela ambientale. Se preferite, si può anche invertire l'ordine dei fattori, ma il prodotto non cambia. Occorre, dunque, una decisione chiara. La mancanza di serenità nel confronto delle parti coinvolte ha portato ad una esasperazione del problema, ben oltre i termini e i contenuti giuridici del Infatti, la decisione, presa durante l'esame della scorsa legge comunitaria per il 2008, di stralciare l'intero articolo, rinviando così la questione die*, non ha risolto il problema, mantenendo aperta la procedura di infrazione per la non corretta trasposizione della direttiva della Comunità europea n. 409 del 1979 nella legge dello Stato n. 157 del 1992. Nel 2006, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2131 contro lo Stato italiano per la mancata o non corretta trasposizione di parti sostanziali della cosiddetta direttiva direttiva uccelli nella citata legge nazionale. Non solo: a questa infrazione, diretta al Governo centrale, se ne sono aggiunte altre tre, provocate da interpretazioni erronee

A fronte di questa insostenibile situazione di incertezza, nel rispetto di posizioni soggettive, tutte degne di considerazione agli occhi del relatore, la Commissione ha privilegiato l'obiettivo di evitare le conseguenze dell'infrazione n. 2131, giunta alla terza fase della procedura prevista dalla Commissione europea, cioè alla Corte di giustizia, quindi alla fase sanzionatoria.

realtà, il relatore aveva tentato l'equilibrismo di un emendamento di compromesso tra due categorie che hanno rivelato ancora una volta una totale incapacità di dialogo: quella dei cosiddetti ambientalisti, ai quali va tutto il rispetto, e quella dei cacciatori, ai quali va data la necessaria considerazione. Ebbene, il tentativo di mediazione e di compromesso è naufragato a fronte di possibili esposizioni a critiche da parte della Commissione europea e, quindi, di un prolungamento della procedura di infrazione. Il relatore, coscientemente e coerentemente, ha ritirato il proprio emendamento di compromesso, e sono stati approvati due emendamenti identici, con il parere favorevole del Governo e del relatore: questo, per verità di cronaca. di cronaca. Pertanto, in base a questi nuovi emendamenti, viene gestita una situazione che potrebbe quasi garantire il blocco della procedura di infrazione ed evitare all'Italia una multa milionaria per la non applicazione di una direttiva. Viene gestito, secondo i dettami della direttiva e in base all'articolo 38, l'arco temporale previsto per il prelievo degli uccelli, e nel contempo si assicura la corretta applicazione della direttiva, richiamando anche la Guida interpretativa della Commissione, che in Italia non era mai stata adottata e che quindi era un ulteriore motivo a sostegno dell'infrazione comunitaria.

Applicando questo articolo e accettando questi emendamenti, l'Italia non fa altro che applicare letteralmente la direttiva europea ed uniformarsi a quanto essa predispone per i Paesi del Mediterraneo.

Il riferimento alla Guida consentirà, inoltre, di interpretare la norma in maniera più stringente da parte delle Regioni ed evitare quelle interpretazioni troppo libere che hanno portato ad ulteriori infrazioni.

con l'unanime consenso della 14ª Commissione e il parere favorevole del Governo, che vieta anche in Italia l'uso di prodotti derivanti dall'uccisione delle foche. L'approvazione di questo emendamento, che ha dato luogo all'articolo 46 del disegno di legge, pone l'Italia in linea con tutti gli altri Paesi europei e rende esecutiva la fase sanzionatoria del regolamento europeo che scatta nel prossimo mese di agosto. Altrettanto delicato è il tema dei rifiuti. Un problema che, nel giudizio della Commissione, ha trovato vasto consenso è il riconoscimento di determinati materiali

dalla classificazione degli stessi come rifiuti: quindi, non più rifiuti ma sottoprodotti, con tutte le analisi scientifiche e tecniche del caso. Si tratta in particolare dell'articolo 19 e dell'articolo 20, che anticipano anticipano alcune disposizioni di attuazione della direttiva sui rifiuti. In tema di agricoltura non vi sono

alla classificazione delle carcasse suine (articolo 25), alla produzione delle uova (articolo 28), all'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta (articolo 30), agli organismi nocivi ai vegetali (articolo 31), altre iniziative che interessano i perfezionamenti nel settore della OCM vino. Per quanto riguarda il delicato campo dei diritti civili, non da ultimo sottolineiamo quegli articoli diretti ad adeguare l'ordinamento nazionale agli standard e alle procedure concernenti la tutela dei diritti civili. In questo contesto figura il recepimento delle decisioni quadro in materia di tutela della vittima nel procedimento penale, di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, di repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (articoli 49 e 51). A tali A tali decisioni quadro si possono aggiungere anche altre normative europee, come la direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare (articolo 48), la direttiva sul pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, o altre direttive, in materia di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, o in materia di fonti energetiche rinnovabili, in materia ambientale, dei trasporti, e molto altro ancora. Altri temi sono stati introdotti, come sempre accade, con gli ultimi emendamenti presentati sia dal Governo, sia da altre fonti, che hanno colmato alcune lacune che esistevano nella legge comunitaria. sincero rammarico per la forzata esclusione di numerosi emendamenti su temi vari, sicuramente innovativi, certamente migliorativi del lavoro che abbiamo fatto in Commissione, ma ritenuti ma ritenuti improponibili in base all'articolo 81 sull'invarianza di bilancio, che la 5a Commissione ha applicato - diciamo con un pizzico di ironia - con grande attenzione e con grande prudenza. sincero dal relatore a tutti i membri della 14ª Commissione, alla presidente Boldi, che ascolteremo fra poco, al personale degli uffici, che ha lavorato con grande impegno e ha portato a termine un lavoro davvero complesso: mettere d'accordo le normative europee, spesso individuate come ostili o comunque contrarie a certe esigenze territoriali, con le idee e le aspirazioni di molti colleghi non è stato facile. Desidero inoltre ringraziare tutti i colleghi che da adesso in poi, con il dibattito e con l'illustrazione dei loro emendamenti, sicuramente renderanno migliore e più ricco questo documento. Vi ringrazio ancora e mi pongo all'ascolto delle vostre proposte. *(Applausi

la partecipazione che il Parlamento deve e può dare, specialmente dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, all'Europa all'Europa e alle due fasi: la fase di formazione della legislazione europea e la fase di recepimento della legislazione europea. Se approverete il testo che vi è stato sottoposto, questa è l'ultima volta che la Relazione sarà approvata con questi contenuti e in questi termini, perché - come è stato già spiegato - ci saranno due relazioni, una a a consuntivo e un'altra che indicherà chiaramente quali sono gli obiettivi del Governo nell'anno a seguire. Credo veramente che ci siano molte novità dal punto di vista procedurale, novità indispensabili per adeguare i lavori parlamentari al Trattato di Lisbona. di Lisbona. So che, specialmente nell'altro ramo del Parlamento, si sta lavorando per una modifica più completa della legge Buttiglione; ma noi abbiamo ritenuto comunque di introdurre delle modifiche, perché questa rielaborazione richiederà giocoforza dei tempi che saranno più lunghi (ci vorrà almeno un anno ancora per arrivare ad una rielaborazione completa), mentre penso che le Aule parlamentari abbiano bisogno di poter lavorare da subito sugli argomenti europei, con le regole nuove che noi abbiamo introdotto. Quando ci sarà la riformulazione e la revisione globale della legge n.

maggiori informazioni, maggiore coinvolgimento e quindi con maggiore possibilità di capire che cosa può rappresentare l'Europa per l'Italia e che cosa possono dare le Camere parlamentari italiane come contributo alla legge europea.

non vorrei disturbare il Ministro. PRESIDENTE.Ministro Ronchi, il presidente D'Alia ha richiamato la sua attenzione.

e le norme contenute nel Trattato con riferimento al rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente di formazione delle norme comunitarie, ci apprestiamo in buona sostanza ad esaminare una disciplina complessa ed eterogenea nelle stessa forme che sono state utilizzate prima della ratifica del Trattato di Lisbona. Tutto questo non va bene, perché non è assolutamente conforme

Siccome l'illustrazione della questione pregiudiziale è propedeutica ad una richiesta di stralcio riguardante le deleghe sul complesso delle norme penali, e siccome credo sia un tema estremamente importante, mi

su tutto il sistema giuridico, e lo ha in maniera ancora più grave e più pesante, senza alcuna garanzia di carattere costituzionale, con riferimento al sistema penale. Siamo garantisti quando ci interessa; quando dobbiamo fare un ragionamento su come viene applicato in Italia il sistema penale comunitario,

pregiudiziale di costituzionalità al nostro esame. Non voglio entrare nel merito, perché non è questa né la sede né l'occasione per affrontare il complesso e il merito delle disposizioni contenute nella legge comunitaria. Mi limito solo a fare un ragionamento riguardante il complesso circuito della formazione e della integrazione nell'ordinamento interno del diritto comunitario.

che non è di mero indirizzo ai Governi, ma un ruolo pregnante nel processo di formazione della normativa comunitaria. Ha attribuito infatti ai Parlamenti nazionali il compito di intervenire anche, attraverso un complesso sistema di corresponsabilità e di verifica dell'attuazione concreta dei cosiddetti principi di sussidiarietà, nella fase in cui il Governo partecipa, in sede di Commissione e di Consiglio, alla formazione della normativa comunitaria. Tutto questo non lo troviamo nel sistema che

definitivamente del ruolo di intervenire nel processo di attuazione della normativa, affidando con delega, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, al Governo il potere di disciplinare normativamente interi settori del nostro ordinamento giuridico, e che questo diventi lo strumento ordinario e permanente attraverso cui si recepisce la normativa comunitaria è certamente sbagliata, al di fuori

di elaborazione delle norme, debbano avere un ruolo attivo e propositivo, anche vincolante, nei confronti degli Esecutivi nazionali e di chi, quindi, andrà poi a definire il complesso delle disposizioni. Se così è - ed è così - è evidente che già ci troviamo di fronte ad un sistema rispetto al quale il Parlamento non ha più alcun ruolo nella produzione delle norme e questo, di per sé, non funziona. Tutto questo poi dà vita ad una serie di distorsioni

estende questa disciplina anche ad Internet, equiparando, sotto ogni profilo, alla disciplina prevista per le concessioni radiotelevisive l'uso, ad esempio, della piattaforma di Internet e della TV che si vede su Internet - si pensi a YouTube - condizionando la possibilità dell'uso di questo mezzo ad una preventiva autorizzazione governativa.

di cui la libertà di manifestazione del pensiero è una parte importante - sia affidato al confronto nella sede esclusiva che la Costituzione ha stabilito, cioè le Aule di questo Parlamento. Questo è il prodotto del modo in cui intendiamo procedere e legiferare in materia comunitaria. Questa è una delle distorsioni più evidenti; ma ve ne è un'altra, che è stata segnalata dall'Unione delle camere penali e che riguarda la circostanza che, con una o più deleghe inserite in questa legge comunitaria - deleghe i cui principi e criteri direttivi sono assolutamente fuori non dalla lettera, ma dallo spirito dell'articolo 76 della Costituzione - si conferisce al Governo il potere di legiferare in materia penale, senza alcun tipo di controllo da parte del Parlamento. Rispetto a questo, credo che, se non vogliamo andare incontro all'ennesima sanzione da parte della Corte costituzionale, queste norme e queste disposizioni - e in tal senso si muove la richiesta che avanziamo oggi in Aula - dovrebbero essere stralciate dal testo relativo alla legge comunitaria. Ciò, perché è evidente che, tanto più è generica e ampia la delega che viene conferita in questa materia, tanto maggiore e discrezionale è il potere del Governo di intervenire sulle norme penali che comprimono i diritti di libertà.

che è totalmente fuori dalla Costituzione, in forza del quale è il Governo, eletto da una determinata maggioranza, che disciplina, senza alcun controllo parlamentare e fuori dalla Costituzione, i diritti di libertà e le sanzioni penali che comprimono questo tipo di diritto di libertà? Ma dove stiamo andando?

di questo modo di intervenire per il recepimento della normativa comunitaria riguarda le procedure di infrazione. Infatti, ogniqualvolta scade una delega e, quindi, si interviene per reiterare il tempo di durata e l'esercizio della stessa, poi si deve intervenire con i decreti correttivi e i testi unici, che non sono meramente compilativi ma conferiscono - anche qui - un potere discrezionale al Governo di legiferare sulla materia: quando tutto questo non avviene, o avviene in contrasto con la normativa comunitaria e con il Trattato, e la Corte di giustizia interviene sanzionando lo Stato italiano, che cosa si fa?

si introducono delle norme che con la normativa comunitaria e la sua attuazione non hanno nulla a che vedere, ma che hanno un'incidenza sull'ordinamento giuridico nazionale.

prioritario ed esclusivo alla 14a Commissione. Quest'ultima non ha - e non dovrebbe comunque avere - il compito proprio delle singole Commissioni di merito, che sono le uniche che possono garantire che il Parlamento esamini il merito delle singole questioni ed eserciti quel controllo che la Costituzione gli attribuisce. per le quali, signor Presidente, a mio avviso non dobbiamo passare all'esame di questo provvedimento, cosa che noi chiediamo con la nostra pregiudiziale di costituzionalità, a garanzia del corretto uso delle regole che presiedono al corretto esercizio del potere legislativo. infatti noi siamo opposizione e domani potremmo essere maggioranza, ma, se passa questo precedente per cui ogni Governo si fa le sue norme penali a suo uso e consumo, dove andremo a finire? In quale Stato di diritto andremo a finire? Questo è il tema di fondo che sottopongo alla vostra attenzione. Nel caso in cui la nostra pregiudiziale non dovesse trovare accoglimento da parte parte del Parlamento, noi riteniamo che le norme penali contenute nelle deleghe debbano comunque essere stralciate, per evitare di accedere ad un pericoloso precedente, che fa a cazzotti non solo con lo Stato di diritto e con la cultura garantista di cui, a volte e a senso unico, ci riempiamo la bocca, ma anche

Si può venir meno sotto questo duplice profilo in diversi modi. Il primo è quello di abbandonare il proprio Gruppo e approdare ad un altro: questo è un modello comportamentale che è stato praticato lungamente all'interno dei Gruppi parlamentari, e sul quale, a mio giudizio, non c'è stata quella censura, né da parte nostra, né da parte della pubblica opinione, che sarebbe stata invece necessaria, anche al fine di recuperare quel minimo di credibilità istituzionale di cui c'è assoluto bisogno. Un secondo modo, sicuramente meno appariscente e meno eclatante, è quello di non intervenire, di accettare in modo silenzioso delle scelte, delle posizioni che non si condividono, che sono contrarie al proprio sentire ed ai propri convincimenti. Proprio per non rientrare con il mio comportamento in questa seconda fattispecie, ho scelto di intervenire per motivare il mio forte dissenso, non tanto rispetto alla legge comunitaria che ci troviamo a discutere, e che a mio giudizio è una sequenza di atti prevalentemente dovuti, quanto rispetto ad un passaggio della Relazione del ministro Ronchi sul quale voglio portare l'attenzione di questa Assemblea. In particolare, nella parte relativa al processo di allargamento dell'Unione europea l'Italia ha sostenuto con piena convinzione le aspirazioni europee di Ankara e prosegue: «Il negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea continua ad essere, in quanto tale, questione controversa all'interno dell'Unione stessa. Da un lato, l'Italia, il Regno Unito, la Svezia e la Spagna sostengono il processo di avvicinamento della Turchia all'Europa, proseguendo con determinazione la loro tradizionale politica di aperto favore per la prospettiva europea di quel Paese; dall'altro lato, si colloca in particolare la Francia, che insiste per la definizione di una forma di partenariato speciale, in alternativa alla piena adesione».

di quella che è la nostra comunità di riferimento. Voglio cercare di affrontare l'argomento ponendo l'attenzione su tre ragionamenti, su tre ambiti e su tre fronti. Il primo riguarda l'appartenenza, o meno, della Turchia all'Europa; il secondo riguarda il pericolo rappresentato dall'Islam; il terzo riguarda, infine, il rispetto che si deve alla pubblica opinione. Per quanto riguarda il primo punto, parto con la risposta dell'editorialista Piero Ostellino a un lettore che chiedeva per quali motivi la Turchia non dovrebbe entrare nell'Unione europea. Piero Ostellino risponde che la principale ragione contraria all'ingresso della Turchia è che la Turchia non è un Paese europeo ma asiatico. Sembra una risposta banale, ma in realtà è una risposta completa, semplice ma definitiva, perché, obiettivamente, la Turchia non è Europa dal punto di vista geografico. Forse qualcuno di voi ha reminiscenze degli studi delle scuole medie superiori: gli atlanti di un tempo qualificavano in maniera certa la Turchia nell'Asia minore,

Forse, se oggi non si condivide il senso di appartenenza all'Europa, è proprio perché mancano questi riferimenti forti a quella che è l'identità e a quelle che sono le radici. Probabilmente, da lì si dovrebbe partire e probabilmente da lì potrebbe rinascere, in qualche modo, il sentimento di appartenenza all'Europa.

le aperture sono possibili solo per Stati appartenenti «chiaramente» al continente europeo, come la Svizzera, la Norvegia e i Paesi dei Balcani. Il *leader* francese non ha precisato il senso di quel "chiaramente", ma sono sottintese le comuni radici geografiche e culturali. e culturali. Papa Ratzinger, poi, ribadisce che "La Turchia è un Paese che non ha radici cristiane ed è permeato, invece, dalla cultura islamica (...) L'identità dell'Europa può essere determinata solo dai contenuti e dalle norme della sua luminosa cultura (...) La Turchia ha rappresentato un continente diverso nella storia e i suoi valori sono diversi, per cui l'adesione sarebbe un grande errore, mentre sarebbe più opportuno offrirle un partenariato privilegiato". Questo è il primo punto. Per quanto concerne il secondo punto, relativo ai pericoli provenienti dall'Islam, l'arcivescovo di Izmir, monsignor Giuseppe Bernardini

Il dominio musulmano è già cominciato con i petrodollari, usati non per creare lavoro nei Paesi poveri del Nord-Africa e del Medio Oriente, ma per costruire moschee e centri culturali islamici nei Paesi d'Europa». Più avanti riporta anche un parere espresso durante un incontro ufficiale da un autorevole esponente musulmano: «Grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo; grazie alle nostre leggi religiose vi domineremo». Forse non tutti hanno la consapevolezza Forse non tutti hanno la consapevolezza del fatto che il primo ministro Erdogan ed il suo partito sono stati ritenuti responsabili dalla Corte costituzionale turca di attività antilaiche per aver tentato di islamizzare la legislazione. Come forse non tutti conoscono

contrari all'ingresso della Turchia nella UE, con un 35 per cento di favorevoli. L'impopolarità della candidatura turca raggiunge il massimo in Austria, con una percentuale dell'80 per cento, circa 24 punti in più rispetto al precedente sondaggio.

danno elementi di riflessione. Non vorrei che passasse anche nell'ambito del centrodestra una logica che non ci appartiene, la logica di tipo leninista; quella logica che abbiamo vista applicata a seguito del sondaggio in Svizzera, dove la popolazione si è espressa contro la costruzione di ulteriori minareti. È quella logica che ci porta a prendere delle posizioni molto diversificate: quando il popolo è in sintonia con il partito, quando è fortemente allineato, allora è maturo e abbiamo la sublimazione della democrazia; quando, viceversa, il popolo si esprime maniera difforme, va in qualche modo indirizzato, educato ed informato. Non è la nostra logica. Per tradizione e scelta siamo rispettosi della volontà popolare, e quando c'è una volontà popolare così forte e così definita dobbiamo necessariamente tenerne conto. Chiudo questo mio intervento ribadendo con forza la mia contrarietà rispetto alle scelte del Governo su questo passaggio specifico. Ripeto, è un passaggio che riguarda esclusivamente la Relazione, nemmeno nemmeno la legge comunitaria, però è l'occasione per esternare il mio pensiero e per farlo conoscere. Approfitto per invitare i colleghi che si sentono di condividere queste osservazioni e che hanno la mia medesima formazione culturale ad intervenire, non dico oggi, ma in tutte le opportune sedi, quelle che riterranno più idonee, per esprimere un parere conseguente. È bene che emerga una voce di dissenso nella nostra parte su questo argomento, perché tacere a mio giudizio è una delle forme nelle quali si possono perdere i propri riferimenti. Ripeto, su questi temi bisogna avere il coraggio di intervenire, di far conoscere il proprio pensiero e, soprattutto, di operare coerentemente rispetto ai propri principi.

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo - che non c'è -, colleghi senatori, nell'intervento che ho consegnato agli atti la prima volta in cui abbiamo affrontato la legge comunitaria in questa legislatura affermavo che l'attuazione del principio contenuto nell'articolo 10 della Carta costituzionale avrebbe potuto diventare uno dei motori per l'armonizzazione della legislazione, tra i vari Paesi e alle mutate condizioni sociali ed economiche. Oltre a ciò, rilevo ora anche un nuovo quadro politico che si va delineando a livello internazionale, dove l'Europa ha un importante ruolo. Il risultato di tale ruolo e del lavoro dell'Unione costituisce un beneficio per i nostri cittadini, non solo se si considera il costo economico del mancato ma anche e soprattutto per la qualificazione che l'ordinamento giuridico nazionale riceve da quello comunitario, che molte volte, però, ci impedisce di di portare avanti i nostri punti politici importanti. Proprio per questo diventa Proprio per questo diventa di stringente attualità il quesito che sollevai allora: cioè, se non si ritenga opportuno addivenire ad una sostanziale modificazione dell'attuale assetto ordinamentale che regge il recepimento delle norme comunitarie nel diritto italiano.

e credo di evidenziare un'esigenza sentita da molti se affermo che sono necessari un intervento e un ruolo diverso da parte dei Parlamenti nazionali nella fase di formazione della legislazione comunitaria. Siamo infatti tutti consapevoli che quando si va a recepire la normativa comunitaria i margini propositivi sono ormai modesti. È nella fase cosiddetta ascendente della normativa dell'Unione che bisognerebbe svolgere un ruolo quanto meno interlocutorio con le istituzioni comunitarie: un nuovo ruolo per tutti i Parlamenti nazionali, e non limitato ai Comitati governativi ristretti, come previsto dal Trattato di Lisbona. È in questa fase che i Parlamenti nazionali possono effettivamente incidere in maniera significativa. Concordo, inoltre, con chi ritiene utile che il Governo - in via

un effettivo e aggiornato monitoraggio nelle varie fasi di concretizzazione di ciascuna direttiva che l'Italia deve introdurre nella propria legislazione. L'articolazione e gli effetti anche sulle legislazioni regionali, oltre che sull'ordinamento propriamente statale, sono innumerevoli e diventa sempre più complesso adeguare a posteriori realtà normative già stratificate. Nel merito, voglio solo soffermarmi sul nuovo principio, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, all'articolo 2, comma 1, lettera *g).* Con tale criterio, unitamente ai due precedenti, si tende all'armonizzazione delle deleghe legislative: nello specifico, si intende stabilire il principio del coinvolgimento delle parti sociali nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive in materia di lavoro e politiche sociali. Ritengo che ci si voglia riferire, in particolare, alla direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, per la cui revisione dovrà essere assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate. Ciò al fine dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi. Il tema del lavoro, così sentito in Europa e ancora più in Italia, richiede sempre di procedere con il consenso di tutti, come ha sempre cercato di fare il nostro Governo. In tempi di crisi, quando il lavoro è minacciato da una situazione internazionale delicata, ciò appare ancora più importante e cogente. Sono certa che il Governo osserverà queste indicazioni non in senso formale, ma chiamando le parti sociali ad un sostanziale impegno, perché la nostra legislazione sia ancora una volta traino ed esempio per tanti Paesi europei che magari si affacciano ora nell'Unione, aspirando ai benefici che ciò comporta, inconsapevoli tuttavia del percorso culturale che sta dietro alle scelte che ci hanno visto antesignani fin dai Trattati di Roma.

retorica. Vorrei esporre il mio ragionamento, a nome del Gruppo ma anche mio personale, come europeista, come federalista europeo convinto,

di rilancio del nazionalismo ma in chiave di copartecipazione alle decisioni. Ciò condurrà ad un Senato degli Stati, che è in coerenza con un'idea federale e federalistica dell'Europa.

prestano grande attenzione, si rendessero conto che, come in passato si diceva che non può darsi il socialismo in un solo Stato, non è oggi pensabile il federalismo in un solo Stato: non è cioè pensabile essere federalisti in un solo Stato senza essere federalisti europei. È questo un ragionamento di coerenza: non si può chiedere un Senato delle Regioni in un solo Stato se non si ha il coraggio di chiedere un'altra Camera, quella che sostanzialmente trasforma l'attuale Consiglio europeo degli Stati in un Senato degli Stati e delle autonomie locali e regionali europee. Se non c'è tale coerenza federalistica anche in Europa, il disegno in un solo Paese non funziona,

di Lisbona - e noi aggiungiamo anche della Carta di Nizza, così fondamentale sui diritti e sui doveri dei cittadini europei - che la legge che la legge comunitaria diventa strumento difficile. Lo diventa anche per motivi interni, perché, nella retorica che accompagna il pensiero unico pre-mercatista, e poi post-mercatista, del ministro Tremonti, la finanziaria *light* genera i mostri del milleproroghe che si allarga e di una legge comunitaria che - stiamo ai dati - ci arriva dalla Camera dei deputati con 12 articoli e ritorna alla Camera dei deputati con 53 articoli. articoli. Già solo questo dato dimostra che tale legge è diventata una sorta di autobus sul quale far salire norme, sulle quali si può anche concordare in linea teorica, ma che in realtà non dovrebbero farne parte per motivi di paletti costituzionali, e regolamentari del nostro Senato della Repubblica, e delle regole che ci siamo dati sulle leggi comunitarie. Alla fine nessuno può essere contrario Alla fine nessuno può essere contrario alle ipotesi delle quali ci troveremo a ragionare, per le quali ci possano essere più finanziamenti europei per una città, per la capitale, o altri emendamenti che vedremo; ma non ha senso inserirli all'interno della legge comunitaria quando è possibile durante tutto l'anno

che mette in difficoltà anche questa legge nel suo complesso, ed è la stessa per la quale la Presidenza del Senato, assieme alla Conferenza dei Capigruppo,

Allora, anche a beneficio del Governo e del ministro Ronchi, cui ho avuto modo in Commissione di dirlo, e affinché rimanga agli atti, voglio ricordare come la soluzione al problema delle infrazioni e delle sanzioni dell'Unione europea non sia quella di inserire tutto l'elenco delle direttive dell'Unione europea, fino a quelle di ieri mattina.

anzi, se non ricordo male, ieri sera, dopo la conclusione della seduta ho ascoltato per caso una conversazione con cui ci si dava appuntamento per la presentazione degli emendamenti del Governo anche con il relatore, il quale è costretto in pochi minuti a conoscere il senso di tali proposte. Ciò dimostra

non notarile) anche un intento programmatico del Governo. Come noto, la presenza in Europa, come la politica estera, non si basa sulle pacche sulle spalle o sull'amicizia personale con questo o quel *leader*; si basa invece sulla continuità con cui siamo presenti ai tavoli europei,

con il disegno di legge n. 1781 il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del provvedimento legislativo, la legge comunitaria annuale, che la cosiddetta legge Buttiglione, cioè la legge n. 11 del 2005 - che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari individua come strumento normativo cardine diretto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario. Il provvedimento affronta i profili relativi alla formazione del diritto comunitario (fase ascendente), al recepimento del diritto comunitario (fase discendente), alla procedura di partecipazione di Regioni,

partecipazione italiana alla formazione del diritto comunitario e sono stati creati nuovi strumenti procedurali per garantire non solo la partecipazione del Parlamento, ma anche delle Regioni e degli enti locali. In secondo luogo, è stato necessario adeguare gli istituti posti dalla legge n. 86 del 1989 alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e, quindi, regolamentare in modo differente i rapporti tra le diverse realtà istituzionali chiamate a partecipare alla definizione del diritto comunitario. Sullo sfondo c'è stata la considerazione del processo di riforma dell'Unione europea, soprattutto per il ruolo di crescente centralità riservato ai Parlamenti nazionali. Il Parlamento italiano ha per molto tempo trascurato la fase ascendente, forse proprio perché non appariva visibile il processo di europeizzazione europeizzazione del nostro ordinamento. Con l'entrata in vigore della legge n. 11 del 2005 (legge Buttiglione) la situazione è cambiata. E ciò in ragione del clima di rinnovato interesse suscitato dall'approvazione del Trattato costituzionale, che tra le sue norme più qualificanti ha previsto proprio il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali. nazionali. L'approvazione della legge comunitaria rappresenta comunque, nonostante le critiche avanzate nel corso dei precedenti interventi, un momento di consapevole partecipazione del Parlamento al processo di integrazione europea. L'importanza di tale passaggio è tanto maggiore se si tiene conto degli appuntamenti istituzionali che attendono l'Unione europea nei prossimi mesi, a partire dalla recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ridisegna l'impalcatura costituzionale dell'Unione europea. Trattato rappresenta una svolta reale per i cittadini del Vecchio continente. È stato abbandonato il Trattato di Nizza, negoziato nel 2000 in Costa Azzurra, fatto per un'Europa a 15 e che necessariamente non teneva conto di tutti gli avvenimenti, anche tragici, accaduti successivamente. Certo, non sarà il nuovo trattato a risolvere i tanti problemi. Ma sicuramente con Lisbona i 500 milioni di europei non rappresentano più solo il mercato unico più importante del pianeta, ma avranno la *chance* di diventare dei *policy makers.* Le nuove norme, infatti, attribuiscono maggiori poteri al Parlamento di Strasburgo, che avrà facoltà di codecisione rispetto al Consiglio europeo. È proprio in quest'ottica che la legge comunitaria deve diventare, non un adempimento burocratico - e questo deve essere l'impegno di tutti noi - ma un provvedimento che costituisce uno dei passaggi di maggiore importanza

in particolare i criteri di ammissibilità e inammissibilità di alcuni emendamenti presentati in Commissione e in Aula. Un punto riguarda il criterio finora utilizzato: infatti, il criterio dell'adeguamento agli obblighi imposti dall'Unione europea è senz'altro giusto allorché la legge comunitaria si pone come l'unico strumento di adeguamento a tali obblighi. Però, se questo strumento non è più l'unico - e abbiamo approvato di recente un decreto-legge che sostituiva la legge comunitaria per le procedure di infrazione - allora bisogna chiedersi se ha ancora senso vincolare la legge comunitaria al rispetto del principio dell'obbligo di adeguamento quando gli altri provvedimenti che danno attuazione al diritto comunitario non soggiacciono a tale tagliola regolamentare. Se poi si considera che la 14a Commissione esamina solo la legge comunitaria in sede referente, ci si accorge che, limitando la sua emendabilità, si rischia di privare la 14a Commissione della possibilità di apportare modifiche importanti

Grazie coerentemente con il principio di effettività, prevede. E, d'altra parte, l'articolo 249 del Trattato di Roma impone agli Stati membri di realizzare il risultato voluto dalle direttive, ma li lascia liberi di perseguire tale risultato con le forme e i mezzi da essi ritenuti più rispondenti. E anche le decisioni quadro, secondo l'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, «salva

lascerebbe preferire un'interpretazione più ampia del concetto di attuazione. Vorrei esprimere la mia soddisfazione, in quanto in Commissione, in sede di discussione e di approvazione di emendamenti, è stato approvato Grazie attribuendo il potere», come previsto nell'articolo 13, così come modificato, «di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico». Si tratta di un emendamento importante; il richiamo all'educazione finanziaria è stato più volte rivolto anche dal Governatore della Banca d'Italia e il mio emendamento - ripeto - andava nella direzione di affermare e rafforzare

Credo che tale disposizione sia molto importante; ricordo che essa è già prevista nel codice di autodisciplina delle società quotate, ma è adottata solo su base volontaria. Inoltre, per garantire la trasparenza dell'attuazione della politica di remunerazione, è previsto che «la relazione

potranno valutare direttamente se i compensi elargiti ai vertici delle società siano commisurati ai risultati ottenuti; quindi si tende a dare ad essi lo strumento per tale valutazione. A mio avviso, è un ulteriore passo avanti

della maggiore importanza e forza che devono avere i Parlamenti nazionali rispetto

quali il Governo e il Parlamento europeo hanno tenuto conto. Mi auguro che si continui su questa strada,

è stato. Infatti, nel tempo ogni provvedimento *omnibus* è stato avvertito come un'occasione da parte del Governo di turno per ottenere deleghe dal Parlamento o, più recentemente, come l'occasione per introdurre emendamenti, strappate la necessità e l'urgenza con il decreto-legge, che hanno costituito vere e proprie mini-riforme di settore. Si tratta di norme rilevanti per importanza e implicazioni, su cui le Commissioni di merito non solo non hanno l'opportunità di intervenire correggendo o integrando l'oggetto della delega o della mini-riforma, a seconda delle circostanze, ma più spesso non hanno neppure la possibilità di discuterne e parlarne. Mi domando, e domando ai colleghi di maggioranza: ma di questo passo, così facendo e così continuando a fare, a che cosa servono che cosa serviranno le Commissioni di merito? Guardate, non è una domanda né retorica né provocatoria, ma solo una richiesta di senso al ruolo che dovremmo essere chiamati a svolgere e che ci vede invece sistematicamente esclusi dall'esercizio della nostra funzione e dalla possibilità di apportare il nostro contributo a provvedimenti importanti e significativi.

per loro natura sono il milleproroghe o la legge comunitaria, appunto) o di quelli che diventano tali - come dicevo - dopo che, come più di recente, i decreti hanno strappato i requisiti di necessità ed urgenza ha finito per collocare la funzione di questo Parlamento in un ruolo improprio rispetto al dettato della nostra Carta costituzionale.

davvero intollerabile, tanto più quando talvolta è utilizzato per deleghe che spesso non vengono necessariamente utilizzate successivamente o che, quando lo sono, vengono talvolta stravolte, come nel caso più recente del decreto legislativo

Come è evidente, quello che sta venendo meno è il principio di trasparenza e di tracciabilità dell'*ite*r parlamentare di approvazione dei provvedimenti, tanto più grave quanto più rilevante è il provvedimento che viene di fatto approvato, per così dire, sotto traccia. Nello specifico e nel merito del provvedimento adesso all'esame dell'Aula, mi riferisco in particolare a due articoli della legge comunitaria che, a mio avviso, avrebbero dovuto avere ben altra considerazione e spazio di trattazione nell'8a Commissione. Si tratta degli articoli 35 e 36, che, presentati come emendamenti, suppongo direttamente dal relatore in 14a Commissione, non hanno consentito il minimo esame in Commissione di merito. Ritengo che l'8a Commissione non sia stata l'unica ad aver subito passivamente l'utilizzo, mi sia consentito, opportunistico della procedura che ho descritto e temo che, in occasione della legge comunitaria, non sia stata neppure la prima volta, lo dico molto francamente. che questo non ci debba indurre a non modificare nel modo più opportuno questa prassi consolidata che, a mio avviso, è assolutamente infelice e inopportuna. Mi sento allora di sollecitare la Presidenza al fine di raccomandare al Governo un uso più equilibrato della facoltà emendativa. Mi risulta infatti che, nella giornata di ieri, si sono aggiunti altri due rilevanti emendamenti del Governo riguardanti il tema delle infrastrutture di trasporto (nello specifico i corridoi TEN, tema certo non banale), e altri sembrano doversi aggiungere nella giornata di oggi (spero di no). In ultimo, vengo davvero al merito degli articoli che ho indicato e segnalo le contraddizioni in essi contenute, ovviamente a mio avviso. L'articolo 35 riguarda alcune norme inerenti ai requisiti di accesso per gli autotrasportatori. Senza entrare nel merito, mi limito ad osservare e a constatare

L'articolo 36 contiene, invece, una norma inerente agli adeguamenti delle tariffe aeroportuali, provvedimento - è bene essere chiari - in sé giusto, visto il lungo tempo da cui non sono state più adeguate e che le configura tra le più basse a livello comunitario, fattore che ha certamente concorso anche alla mancanza di investimenti che si è registrata in questi anni negli scali aeroportuali. Il punto, però, che mi permetto di attenzionare all'Aula e alla Presidenza, anche a futura memoria, dato che questi non saranno temi che lasceremo di certo cadere, concerne la finalizzazione dei proventi derivanti dall'incremento tariffario dei diritti aeroportuali. aeroportuali. In conclusione, pongo alcune questioni. È mai possibile che, a fronte di una destinazione così aleatoria degli investimenti da realizzare, siano solo e soltanto le risorse provenienti dalle tariffe o dalla fiscalità generale a costituire il capitale di rischio per l'impresa, sia essa pubblica o privata, e non anche l'apporto di capitali privati delle stesse società di gestione degli scali aeroportuali? È mai possibile che quando si richiede il ruolo di un'agenzia, di un'*authority* autonoma e indipendente si pensi ormai, nei fatti, ad agenzie governative il cui ruolo di autonomia e indipendenza, come purtroppo anche nel caso dell'ENAC, se non compromesso con la vicenda degli *slot* di Alitalia - e non solo - è di fatto decisamente indebolito? Noi riteniamo che la delega richiesta ed ottenuta nei fatti dal Governo in materia non possa non indurre nella Commissione competente la richiesta di un approfondimento di merito sull'ENAC,

per verificarne l'effettiva rispondenza ai criteri di autonomia e di indipendenza che sono prerogativa essenziale per ogni autorità di vigilanza che si rispetti. infine di segnalare che sulla questione dei diritti aeroportuali forse sarebbe stato più opportuno definire il piano degli aeroporti, commissionato da tempo dai soggetti deputati quali Governo ed ENAC, ma le cui risultanze sono, al di là degli annunci, ancora lettera morta.

e agli effettivi poteri dell'ENAC. Infatti, per esercitare i poteri di autorità di regolazione e controllo occorrono risorse (in particolare umane) di alta professionalità. Attualmente l'ENAC è soggetto ai meccanismi di blocco delle assunzioni a causa dell'ordinamento giuridico di appartenenza (ente pubblico non economico). economico). Ciò comporta che, da un lato, l'ENAC viene chiamato a svolgere complesse istruttorie sul sistema tariffario aeroportuale e, dall'altro, si deve avvalere di limitatissime professionalità con esperienza nel settore della regolazione economica pressoché nulla. Inoltre, non può ricorrere ad *advisor* esterni a causa dei vincoli di spesa determinati dalle varie leggi finanziarie. L'attribuzione all'ENAC del ruolo di autorità di vigilanza in materia tariffaria aeroportuale, così come previsto dalla direttiva comunitaria, comunitaria, lo ripeto, è condivisibile dal punto di vista del principio di ricondurre ad un unico soggetto tutte le competenze in materia di presidio dell'aviazione civile, ma è in palese contrasto con la debolezza strutturale che caratterizza purtroppo l'ente. *(Applausi

Nonostante l'ottimo lavoro della Commissione politiche europee, rimane un pregiudizio fondamentale al provvedimento che ci è stato consegnato dall'Esecutivo: il Governo non ha ancora capito che l'Unione europea, con le sue leggi e le sue istituzioni, non è un fardello che l'Italia deve sopportare, ma una risorsa fondamentale senza la quale il peso internazionale dell'Italia sarebbe inesorabilmente sceso nel contesto mondiale. Una risorsa in termini di legislazione, di finanziamenti economici, che arrivano in Italia con i fondi strutturali, e di apporto culturale dato alla nostra politica. Ma soprattutto l'Europa è un impegno. Un impegno che il popolo italiano ha preso nel 1957, con il Trattato di Roma, quando ha accettato di aderire a valori e principi comunitari, limitando la propria sovranità *ex* articolo 11 della Costituzione. Cari colleghi, tale impegno prevede che gli Esecutivi nazionali adeguino i propri ordinamenti in tutte quelle materie sulle quali l'Unione europea emette norme derivate vincolanti, regolamenti o direttive che siano, per non parlare dei Trattati istitutivi. Non vi è spazio per la discrezionalità e nemmeno per la furbizia. Non si può, cioè, scegliere quali direttive recepire e quali far scadere, e non si può neppure, nel recepimento delle direttive, far finta di adottarne alcune parti e poi tradirne lo spirito di fondo, mantenendo norme italiane correlate con disposizioni in totale difformità. Purtroppo questo Esecutivo ha la brutta abitudine di mettere in pratica entrambi i vizi originali. Ed il Parlamento, nonostante abbia apprezzato davvero sinceramente il tentativo della 14aCommissione e della presidente Boldi di ovviare ad alcune mancanze e di correggere altre storture, non può cambiare l'impostazione di fondo che caratterizza la legge comunitaria licenziata dal Governo. Sull'impianto generale, per ciò che attiene il lavoro della mia Commissione, è da rilevare positivamente il rafforzamento del ruolo del Parlamento nazionale nel processo normativo dell'Unione europea, che è previsto agli articoli 7 e 9 della legge comunitaria. Così come è da apprezzarsi il coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, nonché delle relazioni annuali di attuazione. Anche se, cari colleghi, si deve rilevare che, benché venga previsto l'obbligo di informativa del Governo al Parlamento in merito alle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia, mettendo a disposizione del Parlamento i relativi documenti, questi vengono limitati solo «ai più significativi», solo ad alcune materie (escludendo lavoro ed ambiente, ad esempio), e viene imposto ai parlamentari l'obbligo della segretezza. A noi dell'Italia dei Valori tali limitazioni appaiono come incompatibili con il ruolo del parlamentare, che è quello di rappresentante dei cittadini, e quindi tenuto all'informazione nei loro confronti. Passando all'analisi dei contenuti del provvedimento, di grande significato è stato, sempre per ciò che attiene al lavoro della Commissione, aver recepito la cosiddetta direttiva sanzioni, che impone sanzioni ai datori di lavoro non regolare. I recenti fatti di cronaca - mi riferisco alla bruttissima pagina di Rosarno - hanno mostrato come il fenomeno dell'immigrazione irregolare sia sfruttato dalla criminalità organizzata per avere forza lavoro senza diritti e senza identità. Inserire norme che puniscono questo sfruttamento e che obbligano i datori di lavoro a corrispondere all'immigrato il trattamento economico previsto anche qualora decada il rapporto di lavoro potrà essere uno strumento fondamentale sia per far emergere il lavoro nero che per colpire le cosche che se ne avvalgono. Ritengo rilevante, inoltre, avere previsto una normativa sul trattamento dei rifiuti, poiché la materia è sempre più oggetto di speculazioni e anche di traffici illeciti (vedi il fenomeno delle ecomafie). E pur tuttavia, come dicevo in apertura del mio discorso, colleghi, rimangono nel testo criticità davvero forti e inqualificabili In generale, si potrebbe dire che il Governo appare più solerte a recepire quelle direttive che prorogano i termini entro i quali far entrare in vigore le disposizioni europee piuttosto che le direttive vere e proprie, di merito. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 11, che pospone dal 2008 al 2012 i termini per adottare norme importanti come quella sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. L'Italia dei Valori è fermamente convinta che, per ciò che riguarda la tutela della salute dei lavoratori, non ci possano essere indugi o ritardi, anche in considerazione del già altissimo livello di morti sul lavoro e della fortissima incidenza di patologie legate all'usura o alla mancanza di cautele e precauzioni sul luogo di lavoro. Lo Stato dovrebbe avere fra le sue missioni fondamentali la tutela dei lavoratori esposti ai rischi e ai pericoli, e dovrebbe pertanto adottare un principio di precauzione. Ripetere gli errori fatti nel passato - penso, ad esempio, all'amianto - e disattendere il principio della cautela rispetto agli effetti dei campi elettromagnetici sarebbe un errore imperdonabile. Ed invece l'Esecutivo, appena se ne offre la possibilità, si avvale, purtroppo e sempre, delle proroghe. Insomma, la *ratio* del Governo è di prendere più tempo possibile per adeguare il sistema italiano a quello europeo laddove la politica comunitaria non sia perfettamente corrispondente a quella della maggioranza. Cari colleghi, sinceramente, non sono le disposizioni sui prodotti vinicoli o caseari o sulla combustione delle deiezioni dei volatili che mi preoccupano, anche se queste certamente sortiscono effetti economici ed ambientali che debbono essere valutati attentamente nel rispetto degli operatori economici del settore e dei cittadini che hanno diritto ad un ambiente salubre. Il problema diventa più rilevante in settori che sono stati spesso strumentalizzati dall'Esecutivo e che anche in questo caso continuano ad essere oggetto di speculazione: mi riferisco alla politica dell'immigrazione, a quella del lavoro e a quella sulla fiscalità, che sono parole sconosciute, a volte, ascoltando i commenti della maggioranza. Su questi punti di forte interesse nazionale le criticità ci sono, e sono rilevanti. Mi preme innanzitutto sottolineare come anche in questa legge comunitaria ci sia un grande assente: la direttiva rimpatri, ossia la direttiva n. 115 del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Di questa direttiva soltanto alcune disposizioni sono state recepite dal nostro Governo, attraverso norme come quelle del pacchetto sicurezza che vi si sono ispirate. Queste disposizioni sono tuttavia soltanto quelle che, fra molte presenti nella direttiva, permettevano alla componente xenofoba della maggioranza di portare avanti le demagogiche promesse fatte al suo elettorato. La direttiva n. 115 conteneva infatti anche disposizioni di salvaguardia dei diritti dei migranti, di tutela del trattamento che essi ricevono e di garanzia del loro diritto alla salute e all'asilo, che sono state - immagino volontariamente, e lo sottolineo - ignorate. Il risultato di questa omissione, associata ai respingimenti selvaggi che (anche il cardinal Bagnasco ieri è tornato a criticare) e alla legge Bossi-Fini, di criminalizzare l'immigrazione, emarginandola e facendola finire nel mercato del lavoro nero e, forse, nella devianza, come Rosarno purtroppo ha dimostrato. Altro aspetto problematico è quello relativo ai mezzi di pagamento diversi dai contanti. All'articolo 49 si delega il Governo a recepire la decisione quadro n. 413 del 2001. Orbene, io ed il partito dell'Italia dei Valori siamo certamente favorevoli al fatto che si introducano controlli e sanzioni su chi falsifica tali mezzi di pagamento elettronici o informatici, ma cosa dovremmo dire dei mezzi più ordinari, quelli in contanti, il cui controllo invece è stato abbassato eliminando i tetti massimi che aveva introdotto il ministro Padoa-Schioppa e tutti gli adempimenti legati alla titolarità dei pagamenti? legati alla titolarità dei pagamenti? Forse recepire la decisione quadro potrebbe essere un buono spunto per il Governo per ripristinare i controlli anche sui pagamenti in contanti, ma dubito che nell'ormai conclamata politica del Governo di deregolamentazione dei capitali e di istigazione all'illecito finanziario e fiscale (vedi lo scudo fiscale) si proceda in tale senso. elementi di difformità emergono tra il contenuto della direttiva n. 104 del 2008 e la normativa italiana attualmente vigente, soprattutto in materia di nullità delle clausole dirette a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione, nonché in materia di rappresentanza dei lavoratori circa la salute e la sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di somministrazione. Non potrebbe essere, la direttiva in questione, un buono spunto per procedere ad una riforma del settore e per dare maggiori garanzie a questo mondo sommerso di lavoro senza diritti? di lavoro senza diritti? Cari colleghi, nonostante i rilievi critici che come opposizione attenta e vigile non potevo non porre, ho grande fiducia nel Parlamento, e una convergenza di intenti virtuosa si è già verificata alla Camera, dove molti degli emendamenti dell'Italia dei Valori sono stati accolti, riuscendo ad inserire parte del cosiddetto pacchetto clima nella legge comunitaria. Auspico che lo stesso possa avvenire qua, riuscendo a far sì che si giunga ad una norma che permetta al nostro ordinamento di essere conforme a quello comunitario e non ancora più lontano. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, i lavoratori di molte fabbriche denunciano da tempo il trasferimento delle lavorazioni all'estero, specie in Cina, pratica che si sta rivelando devastante per l'economia del territorio. Al riguardo, c'è ora un primo importante provvedimento, di cui primo firmatario è l'onorevole Reguzzoni, approvato quasi all'unanimità (543 favorevoli e 2 astenuti) alla Camera dei deputati, che introduce l'etichettatura obbligatoria sui prodotti tessili, dell'abbigliamento, dell'arredo casa, delle calzature e della pelletteria. Adesso il disegno di legge è passato all'esame del Senato e le premesse per un risultato positivo sono più che buone. Per la prima volta si stabilisce che nell'etichetta l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. Della denominazione «*made in Italy»* potranno fregiarsi solo prodotti realizzati per almeno due delle fasi di lavorazione sul nostro territorio, mentre per le rimanenti dovrà essere verificabile la tracciabilità. A livello nazionale, i settori interessati a questa legge danno lavoro a circa un milione di persone, ma l'iniziativa è destinata a coinvolgere progressivamente buona parte della produzione nazionale. Basta prodotti di bassa qualità e di dubbia provenienza spacciati come prodotti tipici del nostro Paese! Se noi, rappresentanti della Lega Nord, ne parliamo oggi, in occasione della discussione sulle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza alla Comunità europea, è per fare appello a un voto *bipartisan*, quando sarà il momento, come alla Camera, per presentarci con la massima forza quando sulla questione ci sarà da affrontare l'Europa. La circolazione delle merci è infatti sottoposta alla sovranità comunitaria. E questo è uno dei casi in cui c'è da prendere esempio da Paesi come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, che hanno più volte dimostrato di saper difendere i propri interessi. *(Applausi

come è stato detto dallo stesso relatore, mentre si rafforzano le strutture comunitarie che seguono il progredire del percorso tracciato a Lisbona lento e non secondo il disegno di qualche anno fa, ma è comunque pur sempre il progredire di questo disegno), noi ci presentiamo a questo appuntamento con un anno di

nobilita in qualche modo il carattere routinario dell'esame della legge comunitaria. Mi permetto di dissentire dal giudizio del relatore, perché proprio il quadro

esercitare un ruolo molto più incisivo nel processo di formazione delle decisioni per garantire una base democratica vera e, quindi, un'autorevolezza politica diversa al funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea, attraverso la capacità di dare indirizzi al nostro Governo sulle politiche comunitarie, e a contribuire, settore per settore, alla cosiddetta fase ascendente, cioè alla determinazione delle linee che poi permettono la decisione finale. Come dicevo, in questo quadro è ancora più scandaloso, e non certo consolatorio, il fatto che, primo luogo, ci presentiamo con un anno di ritardo: come la nottola di Minerva, noi spicchiamo il volo al tramonto, quando è già finito tutto, sono già state assunte le decisioni e modificate le direttive. Noi esaminiamo

mi permetto di ricordarlo - di quanto deciso da questa Assemblea all'unanimità, invitando a separare i due momenti per cogliere il senso della specificità dell'atto e la reciproca relazione.

il nostro operare in modo da cominciare a costruire lo spirito di questa modifica che sicuramente ci chiederà un lavoro più lungo.

per dire che abbiamo fatto una buona legge comunitaria, se poi da 12 articoli passiamo a 53 e tutte le volte creiamo questa specie di nebbia,

A seconda del giorno in questo Paese hai dei diritti e dei doveri. Da domani non si sa.

Ministro, colleghe e colleghi, l'esame della legge comunitaria 2009 è anche un occasione per una valutazione della politica europea, in particolare di alcuni suoi recenti sviluppi che suscitano - almeno in me - una viva preoccupazione. Quest'anno la legge comunitaria 2009 prevede delega al Governo per l'attuazione di 31 direttive dell'Unione europea, 7 nell'Allegato A e 24 nell'Allegato B. È più o meno lo stesso numero di direttive da recepire degli anni scorsi, ma devo osservare che man mano che passano gli anni, le direttive dell'Unione europea sono a maglia sempre più stretta. Anzi, alcune direttive emanate nel 2009 sono ormai leggi molto dettagliate. Mi riferisco, ad esempio, alla direttiva 2009/28/CE, emanata il 23 aprile del 2009, sulla promozione delle energie rinnovabili, rinnovabili, che è in sostanza una minuziosa legge in cui i Governi sono trattati come uffici periferici alle dipendenze dell'Unione europea. Non si tratta di un esempio isolato. Il problema è l'atteggiamento radicale assunto dall'Unione europea sulla questione del riscaldamento globale. Come ricordiamo, la svolta della politica europea su questa questione è stata decisa nel Consiglio di primavera dell'8 e 9 marzo del 2007, in cui i Capi di Governo dei 27 Paesi dell'Unione hanno approvato gli ormai famosi obiettivi vincolanti "20-20-20" da conseguire entro il 2020. Aver fissato in termini vincolanti obiettivi molto difficili da conseguire sta inevitabilmente determinando autoritarismo centralistico, tecnocrazia, appesantimento burocratico. Alcuni esempi di questa frenetica e farraginosa attività legislativa e regolamentare europea sulla questione del riscaldamento globale sono il dirigistico ed autoritario regolamento della Commissione n. 244/09 sulla progettazione e produzione delle lampadine per uso domestico, emanato il 18 marzo 2009 (che, tra l'altro, ha messo fuori produzione dal 1° settembre 2009 tutte le lampadine ad opalescenza, prive ancora di decenti sostituti a basso consumo; e ne vedremo delle belle anche qui al Senato); il duro regolamento n. 443/2009 che definisce il livello di prestazione in materia di emissione delle autovetture (vedremo i problemi causati da questo duro regolamento quando entrerà in funzione); il dettagliato piano di lavoro 2009/2011 sulla progettazione e produzione ecocompatibile (documento COM (2008) 660 del 21 ottobre 2008), che prevede la severa regolamentazione di varie decine di gruppi di prodotti; il dettagliatissimo modulo per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili, di cui alla decisione cogente C (2009) 5174 del 30 giugno 2009, una incredibile una incredibile espressione di dirigismo centralistico. Da leggere! Segnalo al riguardo che i regolamenti della Commissione europea sui prodotti che comportano il consumo di energia e che la Commissione europea, al di là del funzionamento autonomo del mercato, si è proposta di rendere ecocompatibili sono decisi dalla Commissione europea senza alcun controllo, né da parte del Parlamento europeo né da parte dei Consigli dei Ministri competenti, sulla base di una semplice delega in bianco contenuta all'articolo 16 della direttiva 2005/32/CE. Devo altresì osservare che, mentre la struttura bipolare dei sistemi politici nazionali rende possibili importanti modificazioni o anche radicali cambiamenti delle leggi nazionali, consentendo sempre l'espressione della sovranità popolare, le direttive europee invece sono sostanzialmente immodificabili da parte dei cittadini. In qualche modo, la struttura non bipolare dell'Unione europea e della Commissione europea costituisce un grosso freno alla dialettica e al confronto ideologico e tende ad impedire la piena espressione politica dei cittadini. Il problema, già grave adesso, sarà sempre più grave in futuro, quanto più l'Unione europea assumerà obiettivi vincolanti ed impegnativi. Il conseguimento di tali obiettivi comporta inevitabilmente autoritarismo e centralismo burocratico. È in sostanza una lesione alla democrazia. Vorrei fare ora una seconda serie di osservazioni. In innumerevoli documenti, la Commissione europea e l'Unione europea hanno mostrato di credere senza il minimo dubbio alla linea di pensiero espressa nei documenti periodici dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) dell'ONU, l'ultimo dei quali è del 2007. In tali documenti, non solamente si ritiene che la causa principale del riscaldamento globale in atto (peraltro finora modesto, limitato com'è a pochi decimi di grado) sia dovuta all'anidride carbonica emessa nell'atmosfera a seguito della combustione dei combustibili fossili, ma si è anche dato credito a catastrofiche previsioni di sviluppo del riscaldamento globale relative a questo secolo (previsioni fatte dall'IPCC e anche espresse in documenti veramente poco scientifici di appoggio, come il Rapporto Stern) e si è infine ritenuto poco efficace l'adattamento delle popolazioni agli eventuali futuri riscaldamenti. Va invece sottolineato con vigore, signor Ministro, che la base scientifica dell'attribuzione del riscaldamento in atto ai gas serra antropogenici è ancora a tutt'oggi piuttosto debole, che i codici di calcolo utilizzati per le previsioni dei futuri sviluppi del riscaldamento non sono affatto sufficientemente affidabili e che le capacità di adattamento dell'uomo ai cambiamenti climatici si sono storicamente sempre dimostrate straordinarie. In sostanza, nella questione estremamente complessa del riscaldamento globale, l'atteggiamento della Commissione europea e dell'Unione europea è stato incredibilmente dogmatico. Per inciso, la mozione approvata in quest'Aula il 1° aprile 2009, in cui veniva rivolto un invito al Governo perché sottolineasse a Bruxelles l'importanza di un molto maggiore affidamento su questa questione alle risultanze della scienza, quella vera, non quella resa succube della politica, non ha avuto alcun seguito. Anzi, continuano ad essere approvati (anche recentemente a Copenaghen) *slogan* propagandistici di basso livello, come quello dell'obiettivo del massimo incremento tollerabile della temperatura media dell'atmosfera terrestre al suolo di due gradi (incremento da misurarsi a partire dai valori di temperatura dei lontani tempi dell'inizio della rivoluzione industriale). Nessuno si preoccupa del fatto che la misura della temperatura media dell'atmosfera terrestre al suolo è assai difficile. Nessun istituto italiano è in grado di effettuare questa misura relativa ad oggi, figurarsi se relativa agli anni passati. In Europa, vi è un solo istituto che dice di essere in grado di effettuare queste misure, ma un recente grave scandalo che lo ha toccato solleva dubbi circa la correttezza di tali misure. Nessuno poi ci dice quale rapporto ci sia tra la concentrazione di gas serra antropogenici nell'atmosfera e il valore della temperatura media dell'atmosfera terrestre al suolo. A ben vedere, questo sbandierato obiettivo dei due gradi centigradi è di difficilissima e questionabile misura e non chiaramente legato ai nostri comportamenti. In sostanza, l'Unione europea guidata da Gordon Brown e Angela Merkel giustifica il perseguimento del valido fine di una maggiore sostenibilità energetica della nostra civiltà tecnologica con i mezzi non corretti della forzatura scientifica, del dogmatismo, della tecnocrazia centralistica, del dirigismo burocratico. Ma, anche in questo caso, il fine non giustifica i mezzi. Questa politica europea, apparentemente così illuminata, sta esponendo l'Unione europea a cospicui pericoli. Ne vedo innanzitutto uno nell'ovvio contenzioso con i Paesi in via di sviluppo, ma ce n'è un altro: è il collasso motivazionale di fiducia nell'Unione europea, se questa si appoggia a basi assolutamente poco credibili.

*(IdV)*. Signora Presidente, colleghi, chiedo ancora una volta che il Governo risponda a numerose interrogazioni parlamentari, presentate nelle sedute nn. 78, 241, 259, 293, 307, 314 e 319, sul ruolo delle autorità vigilanti, in particolar modo della CONSOB, che invece di prevenire truffe e frodi finanziarie e industriali a danno dei risparmiatori e lavoratori va a braccetto con i banchieri e gli imprenditori senza adempiere al proprio mandato di terzietà. Le interrogazioni riguardano il *crac* Freedomland, dove la CONSOB è stata condannata dal tribunale e addirittura ritenuta responsabile della falsità del prospetto, per non aver esercitato la doverosa diligenza: un

scandalosa. Signora Presidente, la prego di sollecitare il Governo. Abbiamo il diritto di ricevere risposte, e non tanto noi, ma quei risparmiatori truffati, quei lavoratori che sono stati messi sul lastrico, in mezzo a una strada. Questi signori, che prendono stipendi e prebende